L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Si fa presente che è in corso la diretta televisiva della RAI che si protrarrà per un'ora. Passiamo dunque alle interrogazioni sull'emergenza alluvione in Piemonte; i senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro per tre minuti ciascuno. Si raccomanda di attenersi rigorosamente ai tempi stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo.

e colleghi, è per me una triste ricorrenza intervenire nuovamente in un'Assemblea legislativa per commentare un evento tragico come quello che si è verificato nella giornata di giovedì 29 maggio in Piemonte. Esprimo profondo cordoglio per i quattro morti causati dalla frana a Villar Pellice. Si è purtroppo trattato di un evento imprevedibile che ci ha lasciati sgomenti per le perdite umane che ha provocato, ma che, stando a tutte le indicazioni ricevute dai tecnici in questi giorni, non è imputabile ad alcuna responsabilità umana. Immediato e tempestivo è stato l'intervento del Governo che ha firmato subito il decreto sullo stato di emergenza in tutta la Regione Piemonte. Ringrazio l'intervento puntuale del sottosegretario Bertolaso con il quale in passato abbiamo avuto modo di di lavorare con importanti risultati sia nella gestione delle emergenze sia nella realizzazione di una rete di protezione civile - colgo l'occasione di ringraziarlo anche per questo - che nella Regione Piemonte rappresenta un modello di riferimento per tutti. Oltre alle cifre stanziate per la prima emergenza per le zone di Torino e Cuneo, che mi auguro vengano incrementate, segnalo anche nel Verbano-Cusio-Ossola il Comune di Trasquera e nel Novarese il comune di Varzo. Mi permetto di segnalare al Governo alcune iniziative di carattere strutturale che evitino di ricorrere all'imposizione fiscale per reperire i fondi necessari ad affrontare il ripristino delle opere pubbliche e la ricollocazione di quelle private: in particolare, i proventi di circa 900 milioni maturati dal bollo bancario imposto dalla legge n. 35 del 1995, soldi che in origine dovevano servire per la ricollocazione delle imprese, che sono però rimasti nel bilancio dello Stato e mai destinati alla Regione Piemonte. Chiediamo, quindi, di adottare una soluzione per provvedere al progressivo ripristino dei fondi non distribuiti. Inoltre, con l'attuazione della legge Bassanini, le Regioni hanno ottenuto il conferimento di nuove funzioni, fra cui la gestione del demanio idrico. Le Regioni avevano chiesto di poter mantenere gli introiti incamerati con la nuova competenza demaniale, ma così non è stato. In pratica, le Regioni sono state gravate dell'onere della gestione del demanio idrico senza avere un riscontro in termini di entrate aggiuntive reali. L'immediata priorità, però, in questo momento, è la pulizia degli alvei intasati dalla piena e per questo chiediamo che venga inserita nell'ordinanza la possibilità di autorizzare rapidamente, senza che i sindaci debbano ricorrere ad aste, la vendita del materiale estratto, estratto, al fine di velocizzare questa pratica assolutamente necessaria. Al Governo chiediamo anche di escludere dal Patto di stabilità le spese cui dovranno far fronte la Regione, le Province ed i Comuni per il ripristino della situazione precedente l'alluvione nelle Province di Torino e di Cuneo. Concludo segnalando, a nome del senatore Barelli, la criticità verificatasi nella Provincia di Roma, in particolare nella valle dell'Aniene. [DELLA Presidente, signori Ministri, colleghe, colleghi, come ricordato ora dal senatore Ghigo, l'alluvione in Piemonte, che ha colpito in particolare le le Province di Torino e di Cuneo ma che avuto delle code anche nelle ultime ore in altre province piemontesi, è legata ad un evento meteorologico oggettivamente eccezionale. Ciò nonostante, credo che questo ennesimo episodio di alluvionale riproponga ancora una volta con urgenza e anche con drammaticità - visto che si è dolorosamente registrata la perdita di quattro vite umane - il problema del dissesto idrogeologico in cui versa gran parte dell'Italia, un problema che rappresenta l'eredità avvelenata di decenni di insufficiente e spesso controproducente governo del territorio, che presenta aspetti particolarmente problematici in una Regione con caratteristiche morfologiche ed idrogeologiche come Io credo che intanto vadano salutate positivamente - e anche su questo concordo con il senatore Ghigo - la rapidità e l'efficacia dimostrate nella gestione dell'emergenza dalle autorità regionali, da quelle locali, dalla Protezione civile, dai Vigili del fuoco, dalle centinaia di volontari che sono stati impegnati, rapidità ed efficacia che certamente hanno contribuito a circoscrivere i danni alle persone. Al tempo stesso, e parlo a nome di tutti i colleghi del Partito Democratico eletti in Piemonte, occorre che il Governo assicuri tempestivamente il necessario sostegno finanziario alla riparazione dei danni diretti dell'alluvione, che ad oggi sono stimabili in almeno 500 milioni di euro. Finora, lo ricordo, il Governo ha deciso uno stanziamento straordinario di 5 milioni Più in generale, credo sia auspicabile che il Governo si dia come priorità, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, il rafforzamento delle politiche di manutenzione e messa in sicurezza del nostro territorio. Da questo punto di vista è un segnale tutt'altro che che incoraggiante che, in mezzo ad innumerevoli tagli a spese non proprio superflue predisposte dal ministro Tremonti a copertura delle misure fiscali, la scure sia caduta anche sui fondi stanziati per il 2008 dal Governo precedente per interventi di difesa del suolo nei piccoli Comuni, cioè in quegli oltre 5.000 Comuni italiani (1.300 solamente in Piemonte) che hanno meno di 5.000 abitanti. La nostra speranza e la nostra richiesta è che l'Esecutivo, signor Ministro,

Presidente, signor Ministro, colleghi, nei giorni scorsi, come è stato già ricordato, il Piemonte, in particolare le valli Chisone, Germanasca, Pellice e Susa, sono state colpite da un'alluvione che ha provocato, oltre ad ingentissimi danni, anche la morte di quattro persone (e mi associo naturalmente al al cordoglio per queste morti). Questa nuova calamità naturale si verifica a quattordici anni dalla precedente alluvione del che, è bene si sappia, vede ancora molte questioni aperte e irrisolte. I danni ammonterebbero, all'incirca, a 500 milioni di euro: 250 milioni di euro stimati per la zona del torinese e altrettanti nella zona del cuneese. la necessità non solo di fronteggiare l'emergenza, ma anche di ripristinare quanto distrutto ed eseguire gli interventi di messa in sicurezza del territorio, che richiederanno molto di più dei 5 milioni di euro stanziati fino ad ora. Chiediamo quindi al Governo di conoscere quali misure intende prendere in proposito e se non ritenga, trattandosi soprattutto di problemi infrastrutturali, di affidare la gestione dell'emergenza e del ripristino e le risorse necessarie direttamente alle amministrazioni provinciali e comunali interessate per competenza territoriale, al fine di abbreviare i tempi e semplificaregli *iter* burocratici,

Signor Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, a partire dalle prime ore del mattino del 29 maggio scorso, il Piemonte è stato interessato da un grave evento alluvionale che ha colpito, principalmente, le Province di Torino e Cuneo.

con fenomeni franosi, smottamenti ed allagamenti che hanno causato la morte di quattro persone, parecchie interruzioni al sistema viario ed alle infrastrutture di servizio, lo sgombero, sia pure solo temporaneo, di alcuni paesi e borgate. Gli enti locali, la Protezione civile e le popolazioni stesse si sono immediatamente attivate sia per dare soccorso a chi era più in difficoltà sia per avviare prime opere di ripristino urgente; a loro va il nostro ringraziamento. I cittadini ancora una volta, però, si sono sentiti insicuri nella loro terra, nelle loro case. Le attività industriali, agricole, artigianali e turistiche sono state gravemente danneggiate. È dunque necessario, una volta per tutte, che vengano impegnate risorse adeguate per interventi strutturali e non tampone; è necessario che si prenda coscienza, una volta per tutte, che i problemi che si determinano non sono delimitabili all'interno dei confini amministrativi di questo o quell'altro Comune ed è pertanto necessaria un'azione di grande unitarietà fra i soggetti responsabili della tutela e del governo del territorio, con interventi di scala temporale e territoriale diversa. Chiedo quindi, a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, quali interventi urgenti il Governo intenda attuare per il superamento dell'emergenza alluvionale in Piemonte, anche in termini di erogazione di contributi alle popolazioni colpite e di sostegno alla ripresa delle attività economiche; quali misure e strumenti, anche di tipo legislativo, intenda porre in essere per avviare scelte rigorose di politica territoriale e di corretto governo del territorio, ridefinendo le competenze operative dei diversi enti, in modo da semplificare e rendere più efficace ed efficiente l'attuazione degli interventi programmati. Chiedo, infine, se intenda destinare nella prossima legge finanziaria adeguate risorse per realizzare interventi strutturali e, in particolare, se intenda procedere all'assegnazione delle risorse stabilite dalla legge n. 35 del 1995, che prevedeva di destinare una parte dell'importo del bollo bancario alle imprese alluvionate da delocalizzare.

l'alluvione si sia abbattuta anche sulla nostra valle, come del resto è già successo in altre occasioni, in quanto i territori alpini sono spesso interessati dagli stessi fenomeni. D'altronde, il Consiglio dei ministri, in data 30 maggio 2008, ha deliberato lo stato di emergenza proprio nei territori del Piemonte e della Valle d'Aosta. Il maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuto sulle Regioni italiane del Nord-Ovest ha devastato anche diverse valli laterali della Valle d'Aosta, in particolare la valle di Rhemes e la valle Savaranche. Siamo di fronte, signor Ministro, a cambiamenti climatici importanti, come dimostrano gli studi effettuati. È ancora fresco in noi il ricordo dell'alluvione del 2000, che causò diverse morti anche in Valle d'Aosta. Ci associamo ovviamente al dolore per la morte che questa volta ha colpito abitanti del Piemonte. Piemonte. Siamo davanti ad eventi straordinari, per cui sembra che gli interventi di emergenza non siano più sufficienti, ma siano necessari invece interventi strutturali. interrogazione, chiedo di sapere quali ulteriori iniziative il Governo intenda al più presto adottare per fronteggiare le prime gravi emergenze dei territori valdostani interessati dal maltempo, stimabili - dalle prime valutazioni - in 35 milioni di euro, e soprattutto, una volta stimata l'esatta entità dei danni causati dalle forti precipitazioni dei giorni scorsi, se non ritenga necessario stanziare ulteriori somme per ripristinare le infrastrutture danneggiate e realizzare le opere di messa in sicurezza delle zone colpite, al fine di evitare che l'ennesima alluvione si trasformi in una sistematica devastazione territoriale di dimensioni irreversibili.

con il Parlamento*. Il Governo ringrazia i senatori intervenuti per la sensibilità dimostrata e coglie l'occasione per testimoniare, ancora una volta, il cordoglio del Governo per le quattro vittime che purtroppo si sono verificate a seguito del grave evento atmosferico. Rispetto ad esso, nonostante la eccezionalità della portata,

Grazie, Torino un centro di raccolta e smistamento delle informazioni. Puntualmente, purtroppo, a partire dalle ore 3 del 29 maggio, le precipitazioni hanno cominciato a diventare sempre più diffuse e si è reso necessario procedere con gli interventi straordinari che, come ricordava senatore Ghigo, sono stati di particolare intensità e hanno visto interessate sul territorio delle Province di Torino e Cuneo fino a 600 unità operative, l'invio di sezioni operative in versione alluvione, mezzi anfibi e macchine movimento terra provenienti, oltre Grazie, urgente è risultato strategico l'invio immediato di elicotteri dei Vigili del fuoco provenienti dai reparti volo di Genova, di Bologna e di Pescara, che hanno operato d'intesa con gli elicotteri del reparto volo di Torino. Questi interventi di prevenzione sono stati

logistici alle squadre operative a terra. Il Comitato operativo nazionale della Protezione civile si è immediatamente riunito, sia a Roma che presso le sedi locali, tutto questo, purtroppo, non è servito - come dicevo prima - ad evitare la morte di quattro persone, è però sicuramente riuscito a contenere e a limitare i danni che con frane ed esondazioni di questo tipo si possono sempre verificare. È stata poi data un'immediata opera di informazione alla popolazione che ne ha consentito la salvaguardia, nonostante l'entità dei fenomeni sia stata mediamente assai significativa e in alcuni casi anche eccezionale.

gli interventi a tutela del territorio, ma deve rilevare, senza voler con questo offrire particolari spunti polemici, che il Dipartimento della protezione civile, negli ultimi anni, aveva insistentemente e documentatamente chiesto interventi all'interno della legge finanziaria che, purtroppo, non è stato possibile stabilire. Per quanto riguarda le richieste successive del senatore Ghigo e della senatrice Boldi circa le deleghe da attribuire agli enti locali, specificamente alle Province ed ai Comuni, come è noto, siamo all'interno di una materia definita di legislazione concorrente dalla legge costituzionale n.

opporrebbe qualora le Regioni interessate, ad esempio il Piemonte, intendessero organizzare il proprio livello di protezione civile anche attraverso apposite deleghe alle strutture provinciali che, in taluni casi, risultano essere già pronte

signor Presidente, ai compiti di prevenzione e tutela del territorio in casi di calamità naturali. Riteniamo tuttavia che con il sostegno di tutto il Parlamento potrà essere meglio avviata un'attività più sistematica di tutela del territorio, che richiederà naturalmente la dotazione di adeguati finanziamenti da parte dello Stato, ma che necessiterà anche la dotazione di adeguati strumenti urbanistici da parte dei Comuni e delle Province interessate. È evidente, infatti, che in Comunità che per loro collocazione morfologica e geologica rischiano di essere purtroppo periodicamente interessate da fenomeni alluvionali di questo tipo solo una migliore tutela del territorio, che potrà essere perseguita adottando gli strumenti urbanistici adeguati da parte degli enti locali, potrà essere favorita. Il Governo, quindi, conviene che non è solo attraverso le misure di prevenzione straordinarie e l'impegno straordinario dei Vigili del fuoco e delle forze della Protezione civile che queste calamità naturali possono essere combattute in zone come quelle del nostro Settentrione d'Italia, che purtroppo sono destinate a dover vivere continuativamente con questi allarmi. Sicuramente il Governo, nell'ambito delle competenze che gli sono state affidate, farà la sua parte.

il signor Ministro ha rappresentato in quest'Aula e anche degli impegni che ha assunto per quanto concerne un ulteriore sforzo di incremento dello stanziamento, che oggi ammonta a 5 miliardi di euro e che, per la gestione della criticità e dell'entità dei danni che si sono verificati, è indubbiamente non sufficiente.

dell'articolo 117 del Titolo V della Costituzione), forse anche le materie che riguardano la tutela del suolo e tutto il comparto urbanistico potrebbero essere oggetto di una valutazione complessiva, proprio per evitare

coinvolge le autorità regionali e locali, il Dipartimento nazionale della protezione civile, il volontariato (che all'interno della protezione civile ha un ruolo decisivo) e i Vigili del fuoco. Ha funzionato bene e ha evitato

sulla vita e sull'economia delle comunità colpite, serve un impegno un po' più stringente da parte del Governo. Non si può rimandare alla finanziaria 2009 lo stanziamento minimo necessario per riparare ai danni diretti dell'alluvione. Tra 5 milioni

le competenze dirette in questa materia, ma il governo del territorio nel suo complesso e le normative urbanistiche, e spero che su tutto questo, nell'attuale legislatura, si riesca a fare qualche passo passo in avanti. Ricordo che da almeno 15 anni il Parlamento non riesce a discutere o comunque a concludere una discussione su una nuova

responsabilizzate, hanno risposto molto bene. Colgo inoltre l'occasione per offrire uno spunto al Governo. Il nostro Paese, per le sue caratteristiche geofisiche, spesso

Ringrazio il Ministro della sua risposta. Mi dichiaro parzialmente soddisfatta. L'Italia dei Valori prende atto delle sue dichiarazioni e degli impegni che ha voluto assumere a nome del Governo e che afferma di voler mantenere. Osservo che rispetto ad alcuni quesiti che le ho posto, in particolare sulla tipologia di interventi legislativi per riordinare il sistema, la sua risposta è stata generica, ma spero ci sia occasione di dibattito e di confronto nel prosieguo della legislatura. L'Italia dei Valori vigilerà affinché le sue dichiarazioni, fatte a nome del Governo, non rimangano di circostanza, ma diventino impegni concreti. Auspichiamo, peraltro, che in questa legislatura non si ponga soltanto una pezza ai danni già prodotti, ma si voglia seriamente seriamente affrontare il tema degli assetti idrogeologici. Signor Ministro (mi permetto di fare questo esempio, forse dissacrante, ma concreto e realistico), in questi giorni, nella Provincia di Torino (la mia Provincia), mentre in una vallata piangevamo quattro vittime innocenti di un corso d'acqua, in un'altra parte del territorio, nel Canavese (un territorio anch'esso messo in difficoltà dalle ingenti piogge), il fiume si rivelava una risorsa, visto che era utilizzato come campo di gara dei campionati del mondo di canoa. Un evento sportivo internazionale di rilevanza turistica e quindi di rilevanza economica per il nostro territorio.

Signor Ministro, mi dichiaro soddisfatto per la sua sensibilità e per la sua tempestività, che sono un buon auspicio per tutta quella normativa a cui lei si appresta a porre mano.

portare a termine quei tanti bei progetti che già abbiamo ascoltato e che ha molto chiari nella sua mente. Parto subito da una dolente nota,

Grazie,

Ministro: da quello che mi risulta, nel 2007 proprio dal capitolo dei diritti per le pari opportunità sarebbero stati sottratti 300.000 euro

Fu uno strappo encomiabile alla regola, frutto dell'impegno delle donne; si trattava di un fondo istituito come prima e rilevante risposta ai dati drammatici sulla violenza contro le donne, che è diventata - come lei sa - la più frequente causa di morte, un vero e proprio allarme sociale. Tra i primi atti del Governo Berlusconi vi è, invece, la cancellazione di quel fondo e la sua destinazione alla copertura dell'abrogazione dell'ICI. La conseguenza di La conseguenza di quell'atto che giudichiamo gravissimo - ma lo sa benissimo - è che vi saranno meno risorse per le donne maltrattate, offese e violentate, per i centri antiviolenza e per la prevenzione. Le chiedo, signora Ministro, se intende adoperarsi perché quel fondo venga reintegrato. Se così non fosse, tante donne, oltre a subire violenza, dovranno soffrire anche per la mancanza di aiuto e di quel sostegno spesso prezioso per dare loro la forza di continuare a vivere. Quelle donne saranno più sole e lei lo sa; le vittime sono 14 milioni

Presidente, Ministro, ho sentito sue precedenti dichiarazioni e so che lei si adopererà a fondo per cercare di portare delle soluzioni al tema della violenza sulle donne che, purtroppo, è assolutamente alla ribalta in questi ultimi giorni.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la violenza nei confronti delle donne, come tutti ormai sappiamo e come le cronache puntualmente ci ricordano, è un male sempre più diffuso del nostro tempo, autentico esempio di un degrado morale e civile cui sta andando incontro la società in cui viviamo. È anche, forse, la parte peggiore di una tendenza che vede emergere sempre più lo sgretolamento dell'idea di famiglia e il sopruso dei più forti nei confronti dei più deboli. È una questione delicata, dolorosa, che andrebbe affrontata con un impegno condiviso, uno sforzo comune e coordinato delle istituzioni, associazioni di volontariato, organizzazioni. Mentre il Governo è impegnato a dimostrare l'improbabile equazione criminalità uguale immigrazione, i dati dell'EURES ci dicono che in Italia un omicidio su quattro viene compiuto in famiglia, tra le mura domestiche. Di questi omicidi, il 70 per cento ha come vittime donne e quasi sempre, salvo casi rarissimi, il colpevole è un conoscente o un congiunto diretto. Una ricerca ISTAT del 2006 mostrava dati allarmanti circa la violenza fisica e sessuale subita dalle donne:

a dimostrazione che questo dramma alberga più nel silenzio della vita privata che non nel clamore mediatico suscitato dai reati compiuti da extracomunitari o immigrati clandestini. Credo che il quadro che abbiamo di fronte sia chiaro. Ecco perché è con sconcerto e rammarico che l'Italia dei Valori e l'intera opposizione hanno appreso del taglio di 20 milioni di euro effettuato per lasciar posto all'eliminazione dell'ICI. Certo, non è una cifra esorbitante se confrontata con altri pesanti e discutibili tagli, come i 400 milioni per l'ambiente o i 353 milioni per il trasporto pubblico locale, ma è indicativa, a nostro avviso, della superficialità e del cinismo con cui il Governo intende metter mano al problema. Quei 20 milioni erano destinati ad un Piano per la prevenzione contro la violenza sulle donne e con consenso unanime del Parlamento erano stati approvati con la legge finanziaria 2008 ed avevano già un preciso impegno di spesa: attivazione di numeri verdi, osservatorio per il monitoraggio delle violenze, campagne di promozione sociale, sostegno alle associazioni territoriali. Niente di tutto questo vedrà la luce. Per questo, ministro Carfagna, chiediamo come intende reagire

mi danno così l'opportunità di chiarire la vicenda relativa al taglio del fondo contro la violenza sulle donne e di anticipare quei provvedimenti che intendo intraprendere per contrastare il dolorosissimo fenomeno della violenza sulle donne. In relazione all'azzeramento del fondo relativo al Piano di contrasto della violenza contro le donne e alle polemiche che ne sono seguite, mi preme sottolineare che il Governo ha ben chiaro quale sia la portata nel nostro Paese del problema in oggetto ed è altrettanto ben chiaro quanto il fenomeno sia in aumento. È peraltro di tutta evidenza che contrastare il fenomeno della violenza contro le donne voglia dire tutelare i minori, spesso spettatori passivi di violenza contro le loro madri. I centri antiviolenza svolgono ed hanno svolto una funzione indiscutibile per aiutare donne e bambini in difficoltà, collaborando attivamente con la magistratura per proteggere le vittime di reati gravissimi, sostenerle ed aiutarle nel processo di recupero di dignità e di serenità della loro vita. Questo Governo intende rispondere con i fatti alle problematiche che affliggono la nostra società; appare sinceramente pretestuoso utilizzare la questione degli tagli imposti dal recente decreto-legge n. 93 del 27 maggio scorso per scatenare polemiche destituite di fondamento. Vi spiego il perché Nessuna sottovalutazione vi è stata in ordine alla gravità e alla portata del fenomeno. Il Dicastero ha anche ben presente l'importanza che i centri di contrasto alla violenza hanno nella vita del nostro Paese e nella tutela dei soggetti deboli, ma, come risulta da recentissimi dati ISTAT sulla violenza ai danni delle donne, soltanto il 2,8 per cento si rivolge a tali centri, che pertanto dovranno essere oggetto di una seria riflessione, ovviamente con gli operatori del settore. Si tratta di un lavoro già avviato dal mio predecessore, che ritengo opportuno e doveroso portare a termine, anche perché risponde alle giuste sollecitazioni provenienti dallo straordinario mondo degli operatori dei centri antiviolenza. Vorrei ricordare agli interroganti che, al fine di promuovere queste politiche, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo, denominato Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Lo stanziamento di tale Fondo, senatrice Franco, non è stato ridotto ed è tale che con esso è possibile realizzare un ampio spettro di politiche per i diritti e le pari opportunità tra cui, naturalmente ed ovviamente, anche azioni di contrasto alla violenza sulle donne. Le risorse del suddetto Fondo sono pari, per il 2008, a 96,8 milioni di euro complessivi (50 milioni di euro del 2008 più l'importo non speso del 2007, pari a 46,8 milioni di euro, che è stato riassegnato al Dipartimento). Le risorse di cui oggi è possibile disporre sono quindi pari a 72 milioni di euro, determinati sottraendo all'ammontare complessivo del Fondo (96,8 milioni) le somme impegnate e da impegnare, rispettivamente pari a 9,2 milioni ed a 11 milioni, per le attività già avviate dal Dipartimento dall'inizio del 2008 a tutt'oggi, nonché le somme accantonate dall'ufficio di ragioneria della Presidenza del Consiglio da gennaio ad oggi per le nuove leggi, pari a 4,6 milioni di euro. di numeri di cui gli interroganti sicuramente saranno a conoscenza, in quanto traduzione puntuale e precisa, senza margini di interpretazione, dell'attività contro la violenza sulle donne posta in essere da chi mi ha preceduto alla guida del Ministero delle pari opportunità. Dato il nuovo clima politico che sembra essersi instaurato in questa legislatura, non è certo mia intenzione innescare polemiche contro chi mi ha preceduto, ma i numeri sono tali tali da permettere un'analisi pacata ed approfondita sulla questione, senza scaricare responsabilità dei recenti fatti di cronaca su chi si è appena insediato al Ministero per le pari opportunità, avviando uno *screening* sulle attività fin qui predisposte per cercare di conservare quanto di buono è stato fatto finora. Ricordo altresì agli interroganti che lo stanziamento da destinare per il 2008 al contrasto alla violenza sessuale di genere potrà quindi essere incrementato con decreto del Ministro per le pari opportunità, rispetto ai 3 milioni di euro previsti dal cosiddetto decreto Pollastrini, nei limiti della complessiva disponibilità di 72 milioni di euro. È una somma notevole che potrà - a mio avviso, dovrà - aggiungere risorse ed attività importanti rispetto a quelle già poste in essere. Credo sia una risposta quantitativa alle tante polemiche di questi giorni sui tagli alle risorse per il contrasto delle violenze sulle donne. I soldi, sia chiaro, ci sono; vanno spesi ovviamente con coscienza e senso di responsabilità. Gli italiani, dalla politica in generale e dal Governo in particolare, chiedono concretezza e risultati immediati. quanto riguarda le azioni di contrasto della violenza sulle donne, verranno presentati nei prossimi Consigli dei ministri due distinti disegni di legge. Il primo di essi, di cui sinteticamente illustrerò i punti salienti, è denominato «Misure contro gli atti persecutori», fenomeno dello *stalking*, che negli ultimi anni è balzato purtroppo agli onori della cronaca e che richiede interventi mirati, in parte già predisposti ma non approvati nella scorsa legislatura. È mia intenzione, e del Governo che qui rappresento, ripartire dalle misure contro lo *stalking* che, con il plauso dell'allora maggioranza e dell'allora opposizione, furono approvate in Commissione giustizia senza mai però approdare in Aula, a causa della chiusura anticipata della XV legislatura. Sarà questa un'importante modifica legislativa, che creerà un'autonoma figura di reato, giustificata dall'inadeguatezza del nostro codice a prevenire, contrastare e punire severamente una condotta sempre più diffusa, anche perché blandamente punita dallo stato attuale della legislazione. Il secondo disegno di legge, dal titolo: «Misure contro la violenza sessuale», verrà presentato prossimamente. Prima di concludere, rispondendo alla domanda della senatrice Poli Bortone, mi preme rilevare che stiamo procedendo ad un'analisi accurata del bilancio che abbiamo trovato in eredità. Da una prima verifica dei capitoli di spesa risulta che, per l'assegnazione dei fondi, sono state privilegiate amministrazioni politicamente in linea con il precedente Governo

(precisamente il 10 aprile 2008, quindi tre giorni prima delle elezioni politiche del 13 e 14 aprile), i fondi stanziati per la Festa del cinema dal Ministero per le pari opportunità sono stati ben 490.000 euro. In conclusione, ritengo di poter rassicurare gli interroganti riguardo alle azioni di contrasto al dolorosissimo fenomeno di cui stiamo trattando. Ritengo che tutte le misure e le iniziative per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, al vaglio del Governo e del Ministero che ho l'onore di rappresentare, non verranno minimamente intaccate dal recente decreto-legge del Governo. *(Applausi

Ringrazio la signora Ministro per le sue risposte; prendiamo atto delle cifre che ha esposto, ma ammetterà che sempre di sottrazione di fondi e di risorse alle politiche per le pari opportunità si tratta e mi chiedo perché

Per quanto riguarda le altre misure, siamo naturalmente disponibili ad un confronto serio e costruttivo sullo *stalking*, visto che siamo stati i primi a proporlo,

di curare e implementare le pari opportunità in questo Paese. Ribadisco che, oltre a provvedimenti di tipo punitivo, è fondamentale che si facciano grandissime campagne per cambiare un certo tipo di mentalità, per insegnare ai nostri ragazzi che le donne vanno rispettate.

e ha fatto distinzione fra vecchio e nuovo Governo. Noi dell'Italia dei Valori riteniamo che il problema debba essere risolto senza tener conto del colore politico di appartenenza, ma attraverso un senso di responsabilità politica istituzionale trasversale.

sia nella passata legislatura che in quella presente, nella speranza che venga accolta nel più breve tempo possibile, a tutela delle donne. Dal momento che siamo alla vigilia della futura manovra di bilancio, potrebbe essere utile che già nella prossima il Governo si impegni a rafforzare gli strumenti utili per le politiche antiviolenza.

finestra"). I Gruppi parlamentari hanno comunicato alla Presidenza la designazione dei propri rappresentanti nella 14a Commissione permanente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 4-*bis*, del Regolamento. La composizione della 14a Commissione permanente sarà pubblicata in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

la Camera dei deputati ha stabilito che la votazione finale del decreto-legge sul trasporto aereo avvenga entro la serata di martedì 10 giugno. Nella stessa giornata di martedì le competenti Commissioni del Senato proseguiranno l'esame del decreto-legge in materia di sicurezza pubblica. Non è, pertanto, possibile iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea, per la prevista seduta di martedì 10 giugno alle ore 17, i due decreti-legge sul trasporto aereo e sulla sicurezza pubblica. Per tali ragioni la seduta pomeridiana di martedì prossimo non avrà luogo. L'Assemblea pertanto tornerà a riunirsi mercoledì 11 giugno, alle ore 10 e alle ore 16,30, con all'ordine del giorno la discussione del decreto-legge in materia di sicurezza pubblica, ove concluso dalle Commissioni competenti. Ulteriori decisioni sui lavori della prossima settimana, con particolare riferimento al decreto-legge sul trasporto aereo, saranno assunte dalla Conferenza dei Capigruppo che si riunirà martedì 10 giugno, alle ore 16.